Al riguardo, segnalo che il Ministro per l'attuazione del programma di Governo ha predisposto un emendamento, in corso di valutazione presso le altre strutture governative competenti, con il quale, al fine di consentire il completamento dell'istruttoria prevista dall'articolo 2,

Naturalmente la mia soddisfazione non si estende all'intenzione che il Governo mi sembra abbia di diluire eccessivamente questa operazione che era stata impostata con molta precisione nella legge finanziaria per il 2008 con due distinte disposizioni, la prima delle quali finalizzata ad individuare criteri, presupposti, condizioni per la soppressione di un numero imprecisato di enti inutili che sappiamo essere ancora esistenti in misura ragguardevole

esposti proprio ieri dal ministro Calderoli, che annuncia una nuova ondata di soppressione di enti inutili quando la norma, che è norma vigente, era stata disposta con con precisione e - credo - anche con efficacia, appunto, dai commi 634 e seguenti dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008. Relativamente invece agli enti già individuati, che costituiscono oggetto

delle competenze, del personale, delle risorse finanziarie e strumentali. Si tratta di un'operazione complessa. Credo che, nel percorso di ammodernamento

la loro sorte occupazionale. Questo numero è destinato ad accrescersi, allorquando - mi auguro - si completerà il percorso di disboscamento di tali enti, che la norma contenuta nella finanziaria intendeva Attendiamo quindi che il Governo adotti provvedimenti concreti su questa materia.

interroganti. La questione più importante è relativa alla scelta di un rimborso costante nel tempo delle minori entrate che deriverebbero ai Comuni. Questa scelta risponde alla necessità di fare riferimento ad un dato oggettivo, quello consolidato, cioè all'impossibilità di prevedere la dinamica delle basi imponibili e delle aliquote

copertura è stata operata attraverso una riduzione di impegni di spesa e una migliore razionalizzazione della spesa pubblica. In particolare, sono state diminuite alcune spese, precedentemente incrementate nell'ultima legge finanziaria e nel decreto-legge cosiddetto milleproroghe,

Non risulta poi, contrariamente a quanto affermano gli interroganti, alcuna disposizione volta a rinviare al 2011 l'introduzione di forme alternative ai trasferimenti erariali per i Comuni.

circa l'utilizzo di alcune voci di copertura del decreto, che ha carattere sostanzialmente temporaneo. Le risorse destinate dal Governo all'estinzione del pagamento dell'ICI sono state momentaneamente prese in prestito, per così dire, dai fondi Fintecna, nell'ottica di realizzare uno degli obiettivi prioritari del programma elettorale. Tale decisione tuttavia non contravviene all'impegno preso dalla nostra coalizione, di realizzare opere infrastrutturali nel Mezzogiorno. Tali risorse, infatti, verranno sicuramente e puntualmente riposizionate non appena saranno pronti gli approfondimenti progettuali e tecnici necessari per l'apertura dei cantieri. In sostanza, si trattava di risorse al momento parcheggiate e non immediatamente pertanto, sono state finalizzate alla copertura complessiva del decreto-legge, ma saranno ripristinate quando i progetti saranno più realisticamente attuabili.

secondo punto riguarda la determinazione degli stanziamenti compensativi - tecnicamente si dice non in termini di cassa ma di competenza - che spettano ai Comuni per effetto dell'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale. Questa, evidentemente, è questione complessa. Faccio presente che, nell'audizione svoltasi alla Camera ieri pomeriggio, l'ANCI ha presentato una documentazione tratta dalla valutazione ISTAT per il 2006

Signora Presidente, onorevoli colleghi, a seguito del rapporto fatto tenere dalla prefettura di Torino sul decesso del cittadino extracomunitario avvenuto all'interno del CPT Brunelleschi è emersa la seguente ricostruzione dei fatti. Alle ore 9,35 del 24 maggio scorso personale dell'ufficio immigrazione della questura di Torino, in servizio all'interno degli uffici del centro, veniva avvisato che in uno dei moduli abitativi siti nella cosiddetta area rossa era deceduto un ospite. Il personale stesso interveniva immediatamente insieme al medico di turno riscontrando che, effettivamente, all'interno dell'area giaceva nel suo letto tale Neji Hassan, sedicente cittadino marocchino, nato a Casablanca il 27 Il medico constatava l'avvenuto decesso alle ore 9,45, riscontrando già da un primo esame, l'assenza di segni di violenza o lesioni. Sul posto giungeva anche il medico legale che, compiuto l'esame sulla salma riferiva che, con ogni probabilità, la morte era dovuta ad una crisi acuta ed improvvisa alle vie respiratorie. Il Neji era ospite del centro di Torino dal 16 maggio, a seguito di trattenimento da parte del questore di Padova. Va precisato che un cittadino tunisino, ospite dell'area, ha affermato di conoscere la famiglia del deceduto ed ha fornito una diversa generalità del defunto, asserendone la nazionalità tunisina. Si tratterebbe di Elmanai Fathi Benali Ben Rihaen, nato il 3 Del fatto è stata data notizia sia all'autorità consolare del Marocco a Torino che all'autorità consolare della Tunisia a Genova. Su disposizione dell'autorità giudiziaria il corpo veniva trasportato all'obitorio cittadino per il necessario accertamento autoptico, che è stato effettuato nella mattina del 27 maggio scorso. Attualmente è stata confermata la circostanza che il cadavere non presentava segni di violenza esterna, ma per la formalizzazione delle risultanze dell'autopsia, che peraltro dovrà accertare l'ora esatta del decesso, si è in attesa dell'esito degli esami istologici e tossicologici, poiché il defunto, dichiaratosi assuntore di eroina al momento dell'ingresso nel centro, era positivo agli oppiacei ed ai metaboliti della benzodiazepina. Conseguentemente era stato sottoposto a terapia metadonica a scalare, terapia effettuata anche nella giornata del 23 maggio. Dalla cartella clinica risulta che lo stesso giorno il defunto era stato visitato e trovato affetto da «flogosi gola più tonsilla sinistra» e che il medico aveva impostato e somministrato la terapia antibiotica ed antipiretica. Le indagini dell'autorità giudiziaria sono volte ad accertare non solo le cause della morte, ma anche le modalità e le circostanze del decesso. In particolare, deve essere chiarito se le condizioni di salute del deceduto si siano aggravate durante la notte e se vi sia stata una richiesta di soccorso, inoltrata dagli altri ospiti del centro, appurando, in caso positivo, i tempi di risposta da parte del personale sanitario presente nella struttura. La procura di Torino ha provveduto ad ascoltare il personale dipendente e alcuni ospiti del centro a conoscenza dei fatti, nonché ad acquisire le registrazioni video effettuate nella struttura. Ritengo doveroso far presente che il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, non appena pervenuta la notizia del decesso, ha disposto un immediato sopralluogo allo scopo di ottenere un quadro conoscitivo completo e preciso. A tal fine, il giorno 27 maggio scorso uno dei direttori centrali dello stesso Dipartimento, accompagnato da funzionari della prefettura e della questura, ha effettuato una visita al centro per accertare, sotto il profilo amministrativo, le circostanze e i fatti occorsi nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 maggio e verificare l'organizzazione e la funzionalità dei servizi erogati dall'ente gestore e la loro corrispondenza alla vigente disciplina. In particolare, il direttore ha sentito il responsabile del centro, il medico coordinatore della struttura sanitaria, i medici intervenuti, compresi quelli del Sert, il responsabile della ASL, una parte del personale della Croce Rossa, i compagni dell'unità abitativa del deceduto. Oltre ai predetti colloqui, è stato svolto un accurato sopralluogo per accertare lo stato dei luoghi ed il livello dei servizi erogati. È emerso che gli ospiti sono risultati di numero molto inferiore rispetto alle potenzialità della struttura: a fronte infatti dei 90 posti disponibili, vi erano 58 persone (55 uomini e 3 donne). L'attività ispettiva ha consentito di appurare che nel centro i servizi assicurati rispondono agli standard qualitativi e quantitativi fissati; infatti, le condizioni di accoglienza dei nuclei abitativi sono risultate confortevoli. Il servizio di assistenza sanitaria, in particolare, è apparso conforme a quanto stabilito nella convenzione con l'ente gestore del centro, essendo garantita, peraltro, la presenza continuativa di personale medico, oltre che paramedico, e la disponibilità di un'ambulanza fissa per eventuali trasferimenti d'urgenza in strutture ospedaliere esterne al centro. Per quanto riguarda poi l'assistenza sanitaria fornita dalle ore 8 del giorno immediatamente precedente il decesso fino al mattino del 24 maggio, giorno in cui è stata accertata la morte del giovane Hassan, è emersa in maniera univoca la presenza ininterrotta di personale medico nel centro, nell'intero arco delle 24 ore. In conclusione, secondo quanto riferito dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, la reale organizzazione del servizio di gestione della struttura, in particolare nei suoi aspetti di assistenza sanitaria, è apparsa pienamente conforme alle regole dettate in materia e riportate nella già citata convenzione. Quanto detto ovviamente senza alcun pregiudizio per l'accertamento - ancora in corso - di eventuali responsabilità di carattere penale, naturalmente rimesso all'autorità giudiziaria. Più in generale informo che il centro Brunelleschi, ove sono avvenuti i fatti, è stato istituito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e il Ministro del tesoro, in data 26 giugno 1998. Esso insiste nell'area dell'ex poligono Genio ferrovieri in corso Brunelleschi, n. 132, nella zona ovest della città. Sotto il profilo della garanzie e della tutela assicurate agli ospiti di tutti i centri, preciso che il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno svolge una costante attività di controllo e vigilanza, in stretto raccordo con i prefetti territorialmente competenti, sulle condizioni di vivibilità esistenti all'interno delle strutture per immigrati, affinché l'intero sistema gestionale sia improntato al rigoroso rispetto degli standard qualitativi e quantitativi indicati nella direttiva generale emanata dal Ministro dell'interno in data 30 agosto 2000 e nelle apposite «Linee guida per la gestione dei centri», approvate con direttiva del Ministro dell'8 gennaio 2003, tese ad assicurare la rispondenza delle modalità di trattenimento alle finalità di necessaria assistenza, anche sul piano sanitario, ed al pieno rispetto della dignità degli stranieri trattenuti. La struttura di Torino è stata oggetto di importanti lavori di riqualificazione e di adeguamento che hanno portato alla installazione, in luogo del preesistente prefabbricato, di moduli abitativi in muratura in grado di garantire condizioni di maggiore funzionalità e vivibilità per gli ospiti. La capienza complessiva del nuovo centro è di 180 posti, suddivisi in due lotti di 90 posti ciascuno. Nello scorso mese di aprile è avvenuta la consegna del primo lotto e in data 14 maggio è stato effettuato il trasferimento degli ospiti nei nuovi locali.

nella convenzione, sulla base dello schema di capitolato unico di appalto per la gestione dei centri di permanenza temporanea ed assistenza e di accoglienza per immigrati irregolari, approvato con decreto del Ministro dell'interno in data 4 aprile 2006, agli ospiti del centro viene assicurato un servizio di assistenza sanitaria. Esso prevede una visita medica al momento dell'ingresso e un primo soccorso sanitario, espletato attraverso apposito ambulatorio inserito all'interno della struttura con presidio medico e personale sanitario ed infermieristico; eventuali trasferimenti, qualora ne ricorra la necessità, presso strutture ospedaliere esterne al centro; la fornitura di medicinali e di presidi sanitari necessari per il primo soccorso e per l'assistenza sanitaria ordinaria; la tenuta di una scheda sanitaria per ciascun ospite. In data 7 giugno 2007 è stato inoltre sottoscritto, ed è operativo, un protocollo d'intesa tra la ASL territorialmente competente, la prefettura, la questura di Torino e l'ente gestore

Signora Presidente, ringrazio il signor Sottosegretario per la risposta che, a nome del Governo, ha voluto dare.

qualcuno si è domandato se questa persona sarebbe morta anche in ospedale. Forse è così, ma la domanda, come lei sa bene, è esattamente questa: perché quella persona non è morta in ospedale?

Ecco, nella parola "ospiti" c'è tutto il carico di ipocrisia - non sua naturalmente, non è un fatto personale - che sta in queste realtà:

le garanzie fondamentali. Sappiamo bene che ci sono stati miglioramenti rispetto alla situazione dei *containers* o delle baracche in lamiera di qualche anno fa, ma nonostante ciò io sostengo, senza tema di essere smentito, che la situazione in quei centri è peggiore

di contenimento delle irregolarità, ma in ogni caso il fatto di sostenere questo non può portarci a chiudere gli occhi e a non vedere che c'è un problema di riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone che in qualsiasi situazione deve essere affrontato, e noi lì siamo in una situazione nella quale questi diritti

su come siamo capaci di affrontare con sincerità tale situazione e di regolamentarla per quello che vale. Infine, un'ultima

che sono alla base dell'interrogazione e della riflessione sollecitata dagli interroganti. Inevitabilmente, dunque, la mia risposta rischia di non essere esaustiva, essa va inserita all'interno di questo lavoro progressivo che è in corso e che continuerà in queste ore proprio per cercare di focalizzare l'attenzione del Governo e delle parti su come sviluppare quelle parole chiave che sono inserite all'interno dell'interrogazione, a partire dal tema della formazione e dell'investimento in formazione. pertanto agli interroganti di tener conto di questo contesto nella valutazione della risposta che mi accingo a dare e che parte proprio dalla legge 3 agosto 2007, n. 123,

costruire la facoltà per gli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale di inserire percorsi formativi interdisciplinari ai fini della promozione e della divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro;

valutare l'effettivo impatto e la concreta operatività della norma, così come costruita, rispetto alle esigenze di sostegno e di accompagnamento dei soggetti che non hanno una particolare capacità finanziaria per realizzare il positivo obiettivo posto dalla norma stessa. In questo momento sono in via di definizione i contenuti e le modalità dei progetti sperimentali di cui all'articolo 4, comma 7, della legge quelli relativi al raccordo tra Ministero del lavoro e della previdenza sociale e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per favorire la conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel confermare nella sua politica prevenzionale il valore strategico della formazione, ha sviluppato un piano di azione rivolto in particolare ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione aziendali e degli addetti. Per quanto concerne l'attività di prevenzione, il decreto legislativo n. 81 del 2008 ha modificato l'assetto istituzionale nell'ottica di una razionalizzazione e di un raccordo tra i soggetti competenti, prevedendo la costituzione, presso il Ministero della salute, del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale organismo ha il compito di stabilire le linee comuni delle politiche nazionali di salute e sicurezza sul lavoro, gli obiettivi e i programmi dell'azione pubblica di miglioramento, nonché la programmazione annuale dell'attività di vigilanza in relazione ai settori prioritari di intervento. Sono stati inoltre rivisitati i compiti della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, individuandola quale sede di confronto tra amministrazioni e parti sociali sulle problematiche di particolare rilievo ai fini della prevenzione. L'INAIL, inoltre, è impegnato, in collaborazione con il Ministero del lavoro e della previdenza per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), alla costruzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in termini di continuità con il progetto «Flussi informativi INAIL, ISPESL, Regioni», del quale l'Istituto è chiamato anche a garantire la gestione tecnica e informatica. La logica che ispira la costituzione di un siffatto sistema informativo è quella secondo la quale, per fare correttamente prevenzione, per promuoverne la cultura e sviluppare le logiche della partecipazione, è necessario ottimizzare la conoscenza del rischio, tenendo conto della peculiarità dei luoghi di lavoro e delle modalità nelle quali si concretizzano gli eventi lesivi. Una conoscenza complessa e progressiva, dunque, patrimonializzata in un organico sistema informativo. In particolare, l'Istituto sta lavorando in termini integrati nella realizzazione del sistema di sorveglianza dei casi mortali, per condividere metodi di acquisizione e sistematizzazione delle informazioni e relazionali tra operatori INAIL, Regioni e servizi di prevenzione delle ASL, per orientare azioni e intervenire nella costituzione di osservatori Per quanto concerne l'ulteriore punto d'interesse evidenziato nell'atto ispettivo, che riguarda la tutela per i soggetti vittime di infortuni sul lavoro, l'eventuale adeguamento della tutela risarcitoria va necessariamente inserito, attraverso la riduzione delle soglie minime previste per l'indennizzo ed una rivalutazione delle indennità economiche, in un contesto più ampio di sostenibilità finanziaria ed in tal senso va approfondito in maniera tempestiva. Con riferimento alle iniziative finalizzate a fornire un'adeguata assistenza ai familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, si evidenzia come l'articolo 1, comma legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro - anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - abbia istituito un apposito fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, conferendo allo stesso la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 2 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 2007, sono state individuate le tipologie dei benefici concessi, nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi. La legge n. 247 del 2007, recante «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale», all'articolo 1, comma 23, ha previsto, in attesa dell'introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi, la destinazione di 50 milioni di euro per l'aumento in via straordinaria dell'indennità per danno biologico. Con specifico riferimento, poi, alla richiesta di notizie circa gli interventi finalizzati a rendere il riconoscimento delle malattie da lavoro meno macchinoso e difficile, si fa presente che è in fase di registrazione presso la Corte dei conti il decreto adottato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della salute, in data 1° aprile 2008, concernente la revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 e 211 del citato Testo unico. Tale decreto amplia l'ambito delle cosiddette malattie professionali tabellate, cioè quelle per le quali opera in favore del lavoratore la presunzione dell'origine professionale della malattia. Ulteriore elemento migliorativo delle nuove tabelle è costituito dall'introduzione di una diversificazione del periodo massimo di indennizzabilità, a partire dalla cessazione della lavorazione di cui trattasi. Precedentemente, infatti, era previsto un periodo unico, pur a fronte di malattie con latenza clinica molto differente. Alla luce delle nuove esigenze, che peraltro impongono un maggior numero di accertamenti e, nel contempo, una maggior incisività degli stessi nella lotta al lavoro sommerso e irregolare, l'INAIL ha comunque avviato la completa informatizzazione del processo di vigilanza, l'integrazione delle procedure di vigilanza con i diversi sottosistemi operativi dell'INAIL (aziende, lavoratori, prevenzione e controllo di gestione), la possibilità di condivisione totale *on line* di ogni informazione con gli altri organismi di controllo, l'istituzione presso la propria direzione centrale rischi di un apposito ufficio di vigilanza assicurativa. Per quanto concerne il profilo inerente la prospettata opportunità di potenziare il corpo ispettivo, vorrei evidenziare che tale potenziamento è stato in realtà già effettuato a seguito delle procedure concorsuali bandite dal Ministero per ispettori tecnici e amministrativi e con l'immissione in servizio dei vincitori e dei concorrenti risultati idonei. Per quanto riguarda, infine, la possibilità di incrementare le risorse umane da adibire a supporto esecutivo degli ispettori del lavoro, sia tecnici sia amministrativi, attraverso la mobilità, si tratta di tematica disciplinata dal Testo unico sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001), rimessa per competenza al Dipartimento della pubblica amministrazione e innovazione, cui è demandata la gestione del personale in disponibilità dipendente dalle amministrazioni dello Stato e dagli egli pubblici non economici nazionali. sicuramente affermare che il Ministero, su questa specifica questione, è disponibile ad una attenta valutazione al fine di giungere ad una ottimizzazione delle risorse presenti. evidente però che una siffatta operazione deve comunque tener conto anche delle peculiarità tecniche di un'attività complessa come quella ispettiva, che richiede specifiche competenze in materia.

anche per la precisazione fatta all'inizio del suo intervento in merito all'incontro, in corso proprio in questo momento presso il Ministero del lavoro, fra le parti sociali per ridefinire l'applicazione del Testo unico sulla sicurezza.

visto che il lavoro rappresenta l'elemento principe del rispetto della vita umana, non può lo stesso lavoro togliere la vita,

e che vuole animare anche il nostro lavoro parlamentare come Partito Democratico e se tale affermazione vale per un territorio come quello della Brianza, a maggior ragione vale per altri territori: pensiamo

signor Sottosegretario, lei ha evidenziato una serie di provvedimenti che sono anche nel segno della continuità rispetto al Testo unico sulla sicurezza approvato nella precedente legislatura. Mi permetto di evidenziarle un aspetto un aspetto che non ho colto nelle sue parole. Lei ha parlato molto di prevenzione e al riguardo il pensiero è comune, è condiviso: la pensiamo allo stesso modo e vogliamo lavorare insieme su questo.

È questo lo spirito che ha animato la nostra interrogazione. Ci auguriamo dunque che il Testo unico venga applicato integralmente e tempestivamente, perché queste morti ci interpellano e noi, con civiltà e umanità, dobbiamo saper rispondere alle vittime. Al tempo stesso - è l'ultimo concetto che intendo esprimere - credo che dobbiamo saper risarcire

cui dovrei partecipare. Cercherò quindi di essere estremamente sintetico, senza sacrificare però la risposta all'interrogazione del senatore Marino. La Molino Cordero Spa di Fossano, in provincia di Cuneo, sulla base delle notizie acquisite presso gli uffici territoriali, presentava originariamente un organico di 24 unità. In seguito al grave incidente, la società è stata trasformata in società in accomandita semplice, nell'intento di scongiurarne il fallimento il quale, invece, come è noto, è stato dichiarato con sentenza depositata il giorno 28 marzo ultimo scorso dal tribunale di Cuneo. In conseguenza dei predetti infortuni mortali, l'INAIL ha provveduto ad istituire, ai sensi dell'articolo 85 30 giugno 1965, n. 1124, recante Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le relative rendite a favore dei superstiti, nelle misure previste al medesimo articolo. In particolare, la rendita viene rapportata al cento per 100 della retribuzione annua percepita dal lavoratore deceduto e spetta al coniuge nella misura del 50 per cento fino a morte o a nuovo matrimonio; a ciascun figlio, nella misura del 20 per cento, fino al raggiungimento della maggiore età ovvero fino a 21 anni se studenti di scuola media o superiore e per tutta la durata del corso, ma non oltre i 26 anni se studenti universitari. In mancanza di coniuge e figli, la rendita spetta agli ascendenti nella misura del 20 per cento se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte; spetta a fratelli e sorelle nella misura del 20 se conviventi con il lavoratore deceduto e a suo carico. Inoltre, come ribadito nell'atto parlamentare, la Regione Piemonte ha approvato una legge per istituire un fondo di solidarietà in favore dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro. Il relativo regolamento di attuazione è stato approvato e sono già state avviate le procedure per la pubblicazione del bando per la presentazione delle relative istanze. L'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto, al fine di fornire un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, l'istituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di un fondo di sostegno, rimettendo la piena operatività dei benefici in parola alla adozione di un decreto ministeriale diretto a definire le tipologie di benefici concessi nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi. Il relativo decreto ministeriale 2 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 2007, prevede l'erogazione a favore dei familiari di vittime di infortuni sui lavoro di una somma *una tantum*, la quale assicuri al nucleo familiare un primo sostegno nei giorni immediatamente successivi al decesso del lavoratore. Viene altresì prevista, nei casi di erogazione del predetto beneficio, la liquidazione, da parte dell'INAIL, di un'anticipazione della rendita di cui al citato articolo 85 del Testo unico. Peraltro, sin dalla pubblicazione del provvedimento è emersa la necessità, dettata da esigenze di giustizia sostanziale, di ammettere al beneficio i familiari delle vittime degli infortuni sul lavoro deceduti nell'intero anno 2007 e non solo i familiari di vittime decedute per infortuni sul lavoro successivamente alla entrata in vigore del citato decreto. Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ha quindi disposto all'articolo 9 che le prestazioni in oggetto vengano erogate «previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale» dall'INAIL e, per gli infortuni del settore marittimo, dall'IPSEMA, e che «in sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a far data dal 1° gennaio 2007». I familiari dei lavoratori deceduti nel grave incidente della Molino Cordero Spa hanno diritto quindi al beneficio in parola, che verrà corrisposto non appena definito il relativo In proposito, aggiungo che già nei prossimi giorni si terranno delle riunioni tecniche volte a definire le concrete modalità di trasferimento delle risorse all'INAIL ed all'IPSEMA e le disposizioni operative per gli uffici.

parzialmente soddisfatto per la risposta. Questa interpellanza nasce da articoli pubblicati sui giornali «La Stampa» e «la Repubblica», i cui titoli riportavano: «Il Molino di Fossano e la strage dimenticata», «Pari dignità per i nostri cinque morti», «I nostri cinque operai morti vittime di serie B per tutti», «Molino Cordero: vittime del lavoro di serie B, dimenticate dallo Stato?». Questo per sottolineare come un tema delicato e importante, come quello delle vittime sul lavoro, troppe volte viene gestito con un'attenzione particolare - a ciò indotti anche dall'attenzione dei *mass media* - nel momento immediatamente successivo all'avvenimento tragico

forse ciò che accade in Provincia pare avere meno dignità di ciò che accade nelle grandi città. Eppure, il problema è assolutamente tragico; ne siamo consci perché nel 2007 abbiamo avuto 1.260 vittime sui luoghi di lavoro; quest'anno, tragicamente, dall'inizio fino ad oggi siamo già arrivati a 488. Sono stati realizzati interventi importanti e significativi, in parte ricordati anche dal Sottosegretario e presenti all'interno dell'interrogazione stessa, sia a livello nazionale sia a livello di Regione Piemonte nella fattispecie specifica, ed è evidente che ancora molto si deve fare. Ciò si evince da un dato semplice: negli ultimi dieci anni abbiamo avuto, per fortuna, una diminuzione del 25 per cento delle morti sul lavoro in Italia; negli stessi dieci anni, in Germania la diminuzione è stata circa del 50

Allora, questa attenzione deve essere trasformata in un'azione continuativa e nella volontà di riflettere affinché i morti vengano considerati tutti uguali. Venerdì 6 giugno si è svolto presso il municipio di Fossano un incontro tra parlamentari, consiglieri regionali della Provincia di Cuneo, la Provincia stessa, il Comune di Fossano, l'Associazione dei familiari delle vittime e gli avvocati, in cui sono stati espressi tre tipi di auspici: in primo luogo, cercare di imporre per legge massimali assicurativi adeguati, per non trovarsi a posteriori a dover piangere su quello che è successo;

in ultimo - ma non meno importante dal punto di vista simbolico - vi è stata una riflessione sulla mancata assegnazione delle Stelle al merito del lavoro alla memoria; questione, richiamata anche all'interno dell'interrogazione, che ha una mera valenza simbolica, ma serve a far far riflettere - visto che è successo anche in altri casi - sul fatto che i morti sono tutti uguali e forse dovremmo porre anche nell'attenzione a posteriori una serie di criteri che vengano dettati dalle nostre coscienze e non dall'attenzione che i *mass media* intendono, di volta in volta, dedicare a ciò che loro ritengono opportuno.

Signora Presidente, l'introduzione di un limite per i neopatentati relativo alla tipologia di veicoli, ed in specie al rapporto tra potenza specifica e tara, era già stato introdotto dal legislatore del nuovo Codice della strada adottato con decreto legislativo n. 285 L'originario articolo 117, al comma 2, prevedeva infatti che per i primi tre anni dal conseguimento della patente non fosse consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica riferita alla tara superiore a 50 kW/t che comunque sviluppino una velocità massima accertata in sede di omologazione del tipo superiore a 150 chilometri orari. Tale disposizione era stata poi abrogata con il decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito in legge 30 maggio 1995 n. 204. Nell'agosto dello scorso anno, il ripetersi di gravi incidenti, occorsi per lo più a giovani alla guida di autoveicoli di cilindrata molto potente, ha indotto il Governodi allora a riproporre l'introduzione di un tale criterio di limitazione per i neopotentati: con il decreto-legge n. 117 del 2007, dunque, si era previsto che per tre anni dalla data di conseguimento della patente (conseguita a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge), ai neopatentati con patente di guida di categoria B fosse impedita la guida di veicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kW/t. Già all'indomani dell'approvazione del decreto-legge, tuttavia, si era palesata una inadeguatezza di tale criterio, specie se applicato in modo assoluto. La norma si dimostrava per taluni profili restrittiva, in quanto il rapporto 50 kW/t escludeva alcune vetture piccole tipicamente ritenute adatte ai neopatentati; per altro profilo, invece, permissiva, in quanto non idonea ad escludere dalla gamma dei veicoli consentiti alcune vetture più potenti, ma anche più pesanti, che erano in grado di raggiungere velocità massima superiore a 180 km/h. Pertanto da subito, sia in sede di conversione del decreto-legge n. 117 del 2007, sia in sede di lavori parlamentari (AC 2480), l'amministrazione dei trasporti ha proposto una riformulazione della stessa disposizione, nel senso di elevare il rapporto potenza/tara a 55 kW/t, ma di coniugare tale criterio con quello di potenza massima consentita non superiore a 70 kW per i veicoli di categoria M1. Tale modifica all'articolo 117, era stata accolta dal Senato nel disegno di legge suindicato. Tuttavia, tale atto non ha potuto concludere il suo *iter* parlamentare per le note vicende della crisi di Governo. Quanto alle sorti del decreto-legge n 117 del 2007, in sede di legge di conversione, il Parlamento non ha inteso accogliere l'emendamento proposto ed ha, al contempo, ridotto ad un anno la durata temporale del limite in parola. Preso atto delle problematiche insorte nel tempo che sono state qui descritte, il nuovo Governo, nel contesto del decreto-legge n. 97 del 3 giugno scorso, su specifica proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha quindi inserito l'articolo 4, comma 4, che prevede una ulteriore proroga, fissata al 1° gennaio 2009, per l'applicazione delle disposizioni attinenti alla limitazione tara/potenza per i neopatentati prevista dall'articolo 117, 2-*bis*, del codice della strada. Sono state accolte, pertanto, le perplessità sollevate da più parti, anche dalle forze dell'ordine, relative all'applicabilità delle norme in questione che avrebbero potuto portare alla conseguenza irrazionale di vietare la guida di automobili di piccola e media grandezza e di alto livello di sicurezza, consentendo invece la guida di vetture meno sicure, più grandi ed impegnative da guidare. Così facendo si consentirà di disporre del tempo necessario per procedere ad una profonda revisione della materia, istituendo un apposito tavolo tecnico per rivedere il parametro relativo al rapporto potenza/peso intorno al quale ruotava la norma relativa ai limiti di guida per i neopatentati.

Come veniva dianzi ricordato, è evidente a tutti, quindi anche a questo Governo, che mi pare lo abbia preso in considerazione, il fatto che il rapporto peso/potenza non sia l'unico elemento di cui tener conto. Questo lo ha ammesso

Com'è noto, lo stato di emergenza ambientale nella Regione Calabria fu dichiarato per la prima volta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 settembre 1997, in relazione ad una situazione di crisi del settore dello smaltimento dei rifiuti non gestibile con poteri di ordinaria amministrazione. Da allora si sono succeduti vari commissari tra Presidenti di Regione e prefetti. In ultimo, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2008, è stato affidato all'attuale commissario delegato il compito di provvedere (in regime ordinario ed in termini di urgenza) al completamento, entro e non oltre il 30 giugno prossimo, di tutte le iniziative ancora di propria competenza già programmate ed in corso di attuazione per il definitivo superamento del contesto di criticità ambientale in atto nel territorio della Regione Calabria. L'attività che i Governi si erano prefissati di svolgere tramite i propri commissari delegati avrebbe dovuto riguardare le specifiche emergenze riscontrate nei settori dei rifiuti, delle bonifiche e della tutela delle acque. Dagli ultimi riscontri a mia conoscenza (sono dati riferiti ad inizio 2007), la gestione finanziaria dell'ufficio del commissario, tra uscite e situazione debitoria, aveva visto registrare la movimentazione di circa 864 milioni di euro. Forse, capire quanto lo strumento utilizzato e le risorse conseguentemente impiegate hanno avuto una loro efficacia non è esercizio puramente retorico. Per ciò che riguarda lo smaltimento dei rifiuti, la situazione attuale, frutto di uno sforzo positivo e concludente, visto la presentazione da parte del commissario delegato di un cosiddetto piano di aggiornamento e rimodulazione del piano regionale dei rifiuti, nonché delimitazione degli ambiti territoriali ottimali dei rifiuti urbani. Ovviamente il nuovo piano, pur registrando alcuni miglioramenti sensibili avviati nell'ultimo triennio, in particolare

Anche per tale motivo le previsioni del piano contengono un cronoprogramma rigidissimo e particolarmente complesso che dovrebbe evitare di incorrere in una gravissima crisi. Se la Regione completasse

se tutto questo fosse realisticamente completato, allora, solo allora, sarebbe comunque indispensabile l'entrata in funzione della nuova linea del termovalorizzatore di Gioia Tauro (o di altro termovalorizzatore) per completare il ciclo dei rifiuti della Regione e poter parlare di gestione ordinaria del settore. Il raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro, la cui realizzazione e gestione è affidata - al solito - a società non calabrese, è attualmente in fase di stallo nonostante le ingenti spese già sostenute per realizzarlo a causa delle proteste che provengono dall'area di Gioia Tauro oggettivamente interessata da varie opere a forte impatto ambientale. Intanto, in Calabria si assiste a una sorta di turismo dei rifiuti che, complici le notevoli distanze da percorrere per giungere in discarica o al termovalorizzatore, finisce per far lievitare le tariffe che i cittadini sono costretti a sostenere. Inoltre - giusto per non farci mancare niente - nelle discariche calabresi trovano posto anche i rifiuti della Campania, non quelli dell'ultimo periodo, in cui i quantitativi scaricati in Calabria sono stati oggettivamente minori e sono serviti in maniera solidale ad alleviare la grave situazione campana, ma le almeno 18.000 tonnellate scaricate tra le discariche di Crotone e Cassano nel 2006. La stessa suddivisione in 14 ambiti e l'iniziale affidamento della raccolta differenziata ad una società mista per ciascuno dei sottoambiti appaiono un elemento di forte inadeguatezza. Si tratta di società sostanzialmente monomandatarie e di modeste dimensioni.

su decisione dell'ufficio del commissario del tempo, con facilitazioni significative e con un sistema che di fatto consegnava alle stesse la reale gestione del settore. Ad oggi, queste imprese del Nord si sono defilate dal mercato calabrese, lasciando una situazione che presenta notevoli appesantimenti non solo sul piano finanziario e gestionale, ma anche e soprattutto su quello delle verifiche giudiziarie in corso rispetto a potenziali fenomeni di infiltrazioni della criminalità organizzata. Tralascio la questione del piano delle bonifiche e del piano delle acque per la brevità che mi sono

per dirla con franchezza, è incredibile che, dopo oltre un decennio di gestione dello Stato nazionale, attraverso l'istituzione dell'ufficio del commissario per l'emergenza ambientale in Calabria, la Regione versi in questa situazione. Il problema è cercare di capire perché non si sia guardato con occhio vigile a quanto stava accadendo.

senza che il commissario conoscesse fisicamente queste persone e senza che esse svolgessero compiti istituzionali. Se tutto questo fosse vero, chiedo di rendere

direttamente, ancorché attraverso delega, intenda contribuire ad affrontare in modo esaustivo le problematiche ambientali della Calabria.

si chiedeva di far luce sulla questione del personale assunto con contratti stipulati dai dirigenti del Ministero dell'ambiente e assegnato all'ufficio del commissariato per l'emergenza ambientale nella Regione Calabria. Mi atterrò dunque soprattutto a questo argomento. Il personale a cui si fa riferimento è quello di cui alle ordinanze di Protezione civile n. 3062 del 6 luglio 2000 e n. 3106 del 20 febbraio 2001, che prevedevano l'utilizzo da parte del Ministero dell'ambiente «per le attività di propria competenza connesse alle situazioni di emergenza e nei suoi limiti temporali» di 15 unità di personale in posizione di comando o di distacco, di 10 esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, nonché, per speciali esigenze, di 20 unità di personale estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato. Veniva altresì stabilito che, nell'ambito delle competenze assegnate al Ministero in relazione all'emergenza ambientale, detto personale doveva essere utilizzato, nella misura del 50 per cento, per le attività relative alla gestione dei rifiuti e bonifiche e, nella misura dell'ulteriore 50 per cento, per le attività riguardanti la tutela delle acque. Appare evidente come le attività poste in essere dal personale previsto dalle citate ordinanze presso la sede del Ministero, pur essendo connesse e funzionali alle situazioni di emergenza, restavano del tutto autonome rispetto a quelle svolte dalla struttura commissariale. È palese, dunque, che spettava al Ministero ogni valutazione non solo sui risultati dell'azione amministrativa svolta, ma anche sull'attività prestata dai dipendenti e sul rapporto costi/rendimenti. Per quanto concerne gli oneri, va precisato che al personale in posizione di comando venivano erogate da parte della struttura commissariale unicamente le somme corrispondenti alle spese per il lavoro straordinario, mentre i relativi oneri stipendiali venivano sopportati direttamente dal Ministero mediante imputazione ai propri competenti capitoli del bilancio. Gli altri oneri, derivanti dall'utilizzo degli esperti e del personale con contratto a tempo determinato, erano sì posti a carico delle risorse assegnate al commissario delegato, ma va sottolineato come il Ministero abbia trasferito sulla contabilità speciale, attraverso le citate e successive ordinanze di Protezione civile, proprie risorse per un importo complessivo di oltre 100 milioni di euro. Si fa inoltre presente che, al fine del contenimento delle spese del personale, il numero dei contratti sottoscritti è stato notevolmente modificato con l'ordinanza n. 3585 del 24 aprile 2007. Il numero complessivo degli esperti e del personale con contratto a tempo determinato veniva ridotto del 50 per cento, passando così da 30 a 15 unità. Si informa anche - è opportuno farlo - che i contratti in parola sono stati sottoscritti dall'Ufficio di Gabinetto e dal direttore generale preposto *pro tempore* alla Direzione generale per la qualità della vita. Con riguardo, poi, all'elenco del personale e ai relativi compensi percepiti per le attività svolte durante il commissariamento, è a disposizione dell'interpellante un elenco completo redatto dalla direzione generale competente. Si rileva, infine, che l'emergenza ambientale nella Regione Calabria si è comunque conclusa il 31 ottobre 2007 e che da questa data si è azzerato l'impiego di personale presso il Ministero sulla base delle citate ordinanze.

di tutte le iniziative ancora di propria competenza, già programmate ed in corso di attuazione, avvalendosi unicamente del personale in servizio presso la struttura commissariale.

gestisce direttamente dei fondi che, invece, sarebbero dovuti servire per affrontare l'emergenza stessa. Stiamo parlando - per capirci - del 2005, quando, cioè, il costo di quel personale era di 700.000 euro